colleghi, come è tristemente noto, nella serata di giovedì 14 luglio a Nizza, a pochi mesi di distanza dalla strage del Bataclan, l'amica Nazione francese è stata nuovamente colpita da un feroce e vile attentato. Il bilancio delle vittime ci consegna le cifre di una autentica carneficina: ottantaquattro morti, oltre duecento feriti, di cui almeno cinquanta in condizioni gravissime; circa una decina i nostri connazionali coinvolti, tra i quali si piangono purtroppo sei vittime. Molte delle persone barbaramente travolte da quel furgone lanciato sulla folla o trafitte dai proiettili sono bambini e adolescenti. Le immagini di quei piccoli corpi straziati sulla strada, con accanto giocattoli o passeggini forzatamente abbandonati, accrescono in tutti noi il dolore e il turbamento per questa assurda strage. A questi innocenti, alla loro infanzia ingiustamente violata e prematuramente interrotta, deve andare il nostro primo pensiero, il nostro abbraccio più forte e la nostra partecipazione più commossa. La ferocia terroristica ha colpito proprio nella notte in cui si sarebbe dovuta celebrare la ricorrenza di un evento emblematico non solo per la storia francese, ma anche per tutte le democrazie avanzate che si ispirano ai valori della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza tra le genti. Tra le vittime vi sono persone di diversa nazionalità, etnia e religione che in quel momento stavano condividendo momenti di gioia e di serena convivialità. Ciò fa assumere all'attentato una valenza simbolica ancora più drammatica perché quelle famiglie, in quel momento, rappresentavano l'unione di popoli e tradizioni diversi, in nome del rispetto reciproco e dei valori condivisi. La strage di Nizza, dopo quelle che hanno funestato il mondo intero, accresce la nostra condanna di fronte a una violenza terroristica incapace di fermarsi persino di fronte all'innocenza di bambini indifesi. Di fronte ad un «terrorismo molecolare», di difficile prevedibilità, in cui un singolo individuo può colpire decine di persone in qualunque momento e in ogni luogo, le istituzioni e le forze politiche devono individuare e attuare ogni strumento utile per la prevenzione e la repressione del terrorismo, per difendere e preservare quei valori di libertà, uguaglianza e fratellanza che sono stati drammaticamente colpiti il 14 luglio scorso. Ciò deve costituire anche un preciso dovere morale per tutti noi, come individui e come cittadini. Il Senato della Repubblica si unisce quindi, con profonda partecipazione, al dolore del popolo francese e delle sue istituzioni, qui rappresentate dall'ambasciatrice di Francia, Catherine Colonna, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza in tribuna. Nel ricordo commosso di chi ha perso la vita, nella vicinanza affettuosa ai feriti e alle famiglie delle vittime, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio e raccoglimento.

in silenzio la commemorazione della strage di

C'è il terrore. Stanno ottenendo quanto volevano e noi stiamo favorendo tutto questo, con un fatalismo che ha dell'incredibile. Non vi è nessun tipo di reazione, prima di tutto in termini culturali. Nel momento in cui abbiamo abbandonato la difesa dei nostri valori e della nostra identità, cosa ci aspettiamo? Noi rispettiamo i valori, l'identità e la religione degli altri, ma è inconcepibile che questi non possano rispettare le nostre. È inconcepibile che si venga qui, come altrove, a cercare di imporre la propria volontà. La difesa dei nostri valori e della nostra cultura cristiana è un dovere di un'Europa che non c'è neanche in questo. Non c'è in questo! Non c'è un insieme, non c'è una polizia unica. Non c'è assolutamente nulla. Si è esposti a tutto. Ma cosa paghiamo oggi? La Francia è il Paese dell'integrazione per eccellenza e sta pagando il prezzo più alto. Ma anche lì - lo dico con serenità, perché d'altronde l'avete visto anche nella reazione della gente a Nizza - la gente è stufa ed è pronta a rinunciare ad alcune libertà per avere un minimo di sicurezza, per non abituarsi a vivere nel terrore. Che facciamo, ci chiudiamo in casa?

una qualunque stazione, di una qualsiasi città d'Italia? Si rende conto di quello che sta accadendo? Si rende conto che così non si può andare avanti, con questo indiscriminato ingresso di tutto e di tutti che avviene ormai da anni? Ne arrivano migliaia al giorno e non siamo in grado di fare nulla. Avete visto che cosa è successo all'isola d'Elba? Accadrà ovunque - l'ho detto più volte - e quando questo problema vi scoppierà in mano la reazione della gente sarà incontrollata. Un Governo e un Parlamento hanno il dovere di guidare questo processo

politica che potrà reggere la rabbia della gente, che non ha colore politico rispetto alle problematiche quotidiane. Dobbiamo ridurci come in Israele, in cui le mamme mandano i figli in pullman diversi a scuola perché almeno ne muore uno solo? Dobbiamo ridurci a questo? Dobbiamo smettere di vivere? Non dobbiamo andare più in un ristorante? I nostri figli o noi stessi: questo vogliamo? O dobbiamo continuare a commemorare - come facciamo oggi - le 84 vittime (per adesso) di Nizza, che sono le ultime di una serie? E speriamo che restino le ultime, ma ho qualche dubbio, perché reazioni vere non ce ne sono. Un'Europa divisa, gli Stati Uniti incerti, è una confusione generale; ci mancava solo la Turchia

Libertà piena per tutto? E per i cristiani cosa c'è? Cosa diciamo? Via il crocefisso? La nostra cultura cristiana la eliminiamo: non più un albero di Natale, perché

però vanno applicate. Non è che l'Italia può diventare il paese di Bengodi dove si viene perché tanto qui non condannano nessuno: così dicono i rumeni, così dicono i georgiani. È incredibile. una presa di coscienza vera e lo dico a chi ci governa e a noi stessi. Guardate quanto accade per le strade, guardate quanto accade nel Paese, non con gli occhi della parte politica, ma con gli occhi del cittadino vero che non ne può più, perché non vede più un vivere civile normale. In questa ottica rivolgo un autentico cominci a reagire oppure ognuno dovrà fare la sua parte. Non costringete tutti a diventare addirittura estremisti per ottenere qualcosa. D'altronde, provvedimento inopportuno rispetto ai temi trattati e a ciò che dobbiamo chiedere alle nostre Forze dell'ordine e di polizia. Non ci può essere alcun dubbio: la gente deve lavorare serenamente in un momento drammatico come questo e noi pensiamo a questo.

Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda i Conservatori e Riformisti, per quel poco che siamo in grado di fare, porteremo avanti una battaglia per preservare la democrazia in questo Paese e i valori cristiani e culturali dell'Italia e dell'Europa.

signor Presidente, la cosa che mi lascia veramente perplesso, anche nello svolgere questo intervento, è il prendere atto, il notare, il considerare come, a partire da alcuni commentatori sulla stampa

a questo sistema di vita, o se preferite, di morte. È la cosa più assurda che possa verificarsi, è la morte politica di un Paese. È la morte stessa delle istituzioni, nel momento in cui ci si abitua

aggiungere qualche argomento perché tutto è già stato detto. Tutto è già stato detto quand'è accaduto a Parigi; tutto è stato già detto per quanto accaduto a Bruxelles; tutto è già stato detto per quanto accaduto a Dacca, per quanto accaduto in ogni circostanza. E noi ancora oggi siamo qui a commemorare e, terminata questa commemorazione, riprenderemo, come se nulla fosse, i lavori del Parlamento, senza avere neppure la considerazione di attribuire la necessaria centralità a questa drammatica situazione, che non è vissuta solo dalla Francia ma che ci appartiene interiormente e intimamente. Presidente, lo chiedo a lei come rappresentante di questa istituzione: è mai possibile

Non possiamo dimenticare che in queste stesse ore in Turchia sta avvenendo un'epurazione che ha come matrice l'integralismo islamico.

ma porta con sé tutto il peso dell'odio e del fanatismo islamico. Come possiamo essere ancora superficiali e non considerare in tutta la sua drammaticità questa situazione? Vede, signor

Ma di cosa vogliamo parlare? Che commemorazione stiamo facendo, se non abbiamo coscienza della situazione che ci sta piombando addosso? È successo ancora una volta, e ancora una volta succederà, perché non siamo coscienti, non siete coscienti di quanto sta accedendo,

signor Presidente, perché gli anni di pace che abbiamo avuto alle spalle sono stati un incidente nella storia e nel percorso dell'umanità. No, Presidente, noi vogliamo che quegli anni di pace continuino anche oggi, ma la pace, come si diceva nell'antichità, deve essere difesa, quando occorre, anche con la spada.

che tali attacchi, perpetrati con feroce determinazione, hanno più volte esposto il fianco a un fraintendimento, all'idea che il disegno terroristico sia figlio anche di tensioni sociali proprie di quel Paese. Questa considerazione ci impedisce di vedere con adeguata lucidità l'altro aspetto, l'altra faccia della medaglia, cioè che il terrorismo di matrice islamista è una ideologia con una caratura che ha tutte le caratteristiche di quelle ideologie che hanno percorso come un vento gelido di morte il nostro Novecento:

che altrimenti dovrebbero diventare un tutt'uno con un giudizio che non trova più riscontro adeguato nella realtà. Su questo invito anche la Sinistra europea, che è sempre stata fondamentale nella lotta contro i terrorismi di varia matrice, a fare un passo avanti, perché solo la considerazione della caratura ideologica di quanto avviene ci può far comprendere come una persona non religiosa, radicalizzata in pochi giorni, sia diventata uno strumento di morte nel giro di un batter di ciglia. Veramente dobbiamo farla questa riflessione, perché le ideologie del Novecento, quelle di matrice occidentale, hanno preso in ostaggio il nome del popolo e nel nome del popolo hanno consumato ogni tipo di eccidio e di strage per molti decenni.

Se non ci sarà consapevolezza adeguata da parte delle nostre istituzioni e dei nostri Paesi, sarà impossibile essere adeguati nel fronteggiare questo scempio. Tuttavia, la seconda considerazione riguarda l'Italia, perché sono 20 gli italiani uccisi dall'ISIS dall'inizio dell'anno e non è possibile che il nostro Parlamento non trovi il modo e il tempo di entrare nel merito di un giudizio corrispondente

e se il nome dell'Italia riecheggia continuamente dietro la rete di complicità che ha fatto sì ci fossero stragi in Belgio come in Francia? Credo che un Parlamento degno di questo nome debba entrare nel merito e debba saper prospettare al proprio Governo adeguate soluzioni e risoluzioni perché si possa fronteggiare una circostanza così difficile. L'ultima considerazione, signor Presidente, è riferita a questo nostro chiacchiericcio, che è meno dignitoso di un silenzio

soprattutto quelle dei più piccoli, travolti sì da un camion, ma forse anche una volta di più dalla stupidità di una certa politica.

alla guida di un camion che ancora adesso si stenta a capire come sia arrivato fino al lungomare di Nizza. Il presidente Hollande, scoraggiato e afflitto dal dolore, quasi ormai incapace di reagire, annuncia a ripetizione che «la Francia è in guerra». guerra». La strage di Nizza di giovedì scorso ha segnato probabilmente un punto di non ritorno nella storia recente della guerra che il terrorismo islamico ha dichiarato alla civiltà occidentale, ormai dall'attentato alle Torri gemelle in poi. A Nizza abbiamo constatato che non sono soltanto i cosiddetti obiettivi sensibili ad essere sotto scacco, ovvero stazioni, aeroporti, centri di potere e monumenti rappresentativi, ma ogni luogo dove è facile raggiungere il maggior numero di persone possibile; dove lasciare un segno indelebile, una macchia di sangue che sarà difficile dimenticare chissà per quanti decenni. E non sono servite bombe, né particolari equipaggiamenti di armi da fuoco, ma è bastato un mezzo pesante, un camion, per portare a compimento una carneficina, che forse mai ci saremmo aspettati, proprio per le modalità con cui è stata perpetrata. Dinanzi a tali atti, occorre mettere in campo misure forti per salvaguardare i propri cittadini, le rispettive istituzioni e quelle sovranazionali. Non bisogna certo essere degli esperti di *security* per capire che negli ultimi tempi Francia e Belgio non si sono particolarmente distinti sotto questo aspetto. In un giorno come il 14 luglio per i francesi gli occhi della sicurezza dovevano essere molto più vigili ed accorti. Mi chiedo e vi chiedo: chi si deve occupare delle nostre vite è in grado di farlo? Ha tutti gli elementi, le competenze e i mezzi per salvare le nostre vite e quelle dei nostri figli? Questo è l'interrogativo a cui qualcuno, di dovere e di spettanza, deve dare una risposta soddisfacente quanto prima. L'osservazione da parte degli organi deputati di singoli individui o di gruppi che si ritiene debbano essere attenzionati, così come il controllo dei flussi migratori o il rafforzamento delle misure di sicurezza in luoghi ritenuti potenzialmente a rischio, si sono rivelati strumenti, per quanto necessari, insufficienti. Accanto a tutte le misure più convenzionali, come ad esempio l'ulteriore rafforzamento della cooperazione internazionale in campo di *intelligence*, abbiamo bisogno di una rivoluzione valoriale e culturale, che argini ogni forma di fanatismo. Dobbiamo promuovere, fin dalle scuole dell'obbligo, un'idea di integrazione e di condivisione di valori comuni più convincente. I bambini di ogni religione e razza devono imparare a rispettarsi e a condividere dei principi laici comuni in cui credere ed in cui rivedersi. Credo che il primo passo verso la normalizzazione della convivenza tra occidentali ed arabi passi per il potenziamento di questa visione laica e valoriale della problematica sociale. La promozione di iniziative condivise comuni su temi storici che ci vedono uniti rappresenterebbe un viatico importante per cercare di avvicinare due mondi che in questo momento sembrano avere davvero pochi punti di vicinanza. I drammatici fatti di Nizza impongono la necessità che tutte le democrazie occidentali e gli Stati di diritto rafforzino la propria coesione in campo internazionale per arginare l'*escalation* terroristica. In gioco c'è il mondo libero, quotidianamente minacciato dal fanatismo terroristico al quale, un dato è certo, non possiamo in alcun modo piegarci. Ciò che abbiamo faticosamente costruito in tanti anni di battaglie civili e di diritto, nel giro di poco sembra sgretolarsi sotto i colpi, i fendenti sempre più perfidi dei portatori di morte che esibiscono il vessillo nero. In Europa, che negli ultimi mesi è stato il fulcro degli attacchi terroristici, quale migliore risposta, se non quella di dimostrare la propria coesione e di riaffermare con forza i propri valori, così da porsi quale capofila di tutti Paesi che si oppongono all'ISIS? Dopo la Brexit, i cui effetti temo si paleseranno solo tra diversi mesi, credo che l'unità politica di tutta l'Unione rappresenti la risposta più ferma ed efficace che si possa dare ad un nemico tanto subdolo. Soltanto un'unità concreta, una collaborazione internazionale senza precedenti, una reale comunione di intenti ed una reazione univoca e decisa di tutti i Paesi europei potranno tentare di arginare l'azione di quanti, costringendoci nel terrore, vogliono di fatto sovvertire le nostre istituzioni, che sono la sostanza stessa della democrazia e della civiltà, e non solo quelle europee. *(Applausi

e che è stata ribadita ieri sul piano parlamentare nella riunione del Governo con i Gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione e nel vertice europeo richiesto dalla Francia dopo l'attentato di Nizza. Sappiamo come l'attacco del terrorismo globale abbia una sua identità culturale. Bernard-Henri Lévy ha definito il fenomeno come: «l'influenza senza contatto, attraverso il contagio e la suggestione fulminea». L'estremismo radicale ne è la dimensione fondamentale e le reti globali di comunicazione sono state utilizzate per l'evoluzione di un terrorismo diffuso e di massa. Cellule e soggetti individuali possono essere autonomi e e non affiliati: si sono radicalizzati via *web* o sono interni al califfato. Sappiamo come i terroristi possono ricorrere a tecniche e risorse Siamo consapevoli che tali soggetti abbiano un dato strategico comune: la nostra civiltà occidentale; la nostra cultura e il nostro modo di vivere. Sappiamo che i terroristi hanno deciso di colpire le comunità civili europee nella loro quotidianità,

europee un ruolo non così passivo nei confronti del jihadismo, se vogliono vivere con noi, perché anche loro devono difendere assieme a noi i valori comuni. Sappiamo, infine, e ribadiamo, insieme al Governo, come nel lungo termine comunicazione e cultura siano fattori strategici nel chiarire senza riserve e senza paure che non sia accettabile la tolleranza nei confronti dell'intolleranza e del fanatismo islamico. Nel contempo, occorre essere capaci di risposte condivise e comuni sotto il profilo sopranazionale, in primo luogo tra i Paesi europei, ma anche coinvolgendo la Russia e gli Stati Uniti. Solo così possiamo vincere la sfida contro gli attacchi terroristici e il populismo crescente che mette a dura prova tutte le nostre conquiste civili ed economiche degli ultimi secoli. *(Applausi Presidente, purtroppo nel giro di pochi giorni due eventi politici tragici e sconvolgenti si sono abbattuti sulla Francia prima e sulla Turchia poi e, più in generale, su tutta l'Europa e anche sul nostro Paese. Anche l'Italia, come è stato ricordato, è stata colpita direttamente con sei vittime identificate.

è stata colpita anche in quanto Paese esposto, come tutti, al rischio che tragedie come questa possano verificarsi anche da noi. L'attentato di Nizza, per le sue dimensioni e modalità, in gran parte ancora oscure, costituisce una novità, sia pur prevedibile e purtroppo prevista nel quadro sanguinario del terrorismo in Europa. Per questo motivo tale attentato ha destato una paura diffusa, persino superiore a quella suscitata dai precedenti attentati. È davvero comprensibile che questo terrorismo, che potremmo definire fai da te te e che non ha bisogno di organizzazioni particolarmente complesse, sia considerato ancora più temibile delle altre modalità del terrore. Vuol dire davvero che il pericolo può arrivare all'improvviso da chiunque e finanche l'inquilino della porta accanto può rivelarsi una minaccia mortale. È ovviamente chiaro a tutti che prevenire fatti del genere è ancora più difficile che fermare, con operazioni di *intelligence*, i gruppi terroristici più strutturati. Presidente, è davvero inutile nascondersi che questa paura diffusa può prestarsi a facili strumentalizzazioni politiche e gonfiare le vele della xenofobia e dei peggiori istinti securitari, diffondendo l'illusione che, per questa via, sia possibile garantire maggiore sicurezza. sicurezza. Noi crediamo che questa è la reale portata della sfida che oggi l'Europa ha davanti: sconfiggere il terrorismo e restituire sicurezza ai cittadini, senza sacrificare la propria cultura e la propria civiltà. di una di quelle grande sfide storiche con cui ogni generazione deve prima o poi misurarsi. In queste occasioni epocali spunta sempre la tentazione di imboccare le strade apparentemente più facili, quelle più sbrigative e rassicuranti, ma è soltanto un'illusione ottica. Imboccare quella strada non soltanto sarebbe eticamente sbagliato, ma significherebbe anche scendere esattamente sul terreno che il terrorismo vuole imporci. Noi dobbiamo invece mettere in opera tutte le misure di sicurezza e prevenzione, è possibile fare solo con un livello massimo di integrazione e cooperazione tra i servizi di *intelligence* di tutti i Paesi. Dobbiamo disporre di forze capaci di intervenire con tempestività ancor più di quanto, purtroppo, è stato fatto troppe volte negli ultimi mesi. Allo stesso tempo, però, dobbiamo sapere che non potremo smarrire per un attimo i valori, le libertà e i diritti democratici che abbiamo conosciuto e costruito in tutti questi anni per tutti. Dobbiamo contrastare e reprimere i canali che portano alla radicalizzazione e attrezzarci per contrastare la propaganda jihadista laddove essa esercita i propri micidiali effetti (quindi, anche sui mezzi di comunicazione), ma - allo stesso tempo - dobbiamo capire perché si è determinata quella radicalizzazione e come identificarla e disinnescarla. In Turchia, poche ore dopo la strage di Nizza, abbiamo assistito a un colpo di Stato fallito e, come è stato efficacemente definito, a un contro-*golpe* riuscito.

l'imprigionamento dei giudici costituzionali che avevano osato opporsi a Erdogan, il tentativo di usare l'alibi del terrorismo per ripristinare la pena di morte, il divieto di espatrio per i funzionari pubblici e addirittura

D'ora in poi saremo alle prese con una Turchia ancora meno democratica di quel che era (e già si trattava di una democrazia più che monca). Anche in questo caso, signor Presidente, c'è davvero una tentazione facile a cui l'Europa e l'Italia debbono sottrarsi, cioè quella del cinismo spacciato per *Realpolitik*. Bisogna usare tutti i mezzi pacifici possibili per difendere i diritti dei cittadini turchi non si può davvero considerare plausibile l'ingresso nell'Unione europea di un Paese che non garantisce più nemmeno il livello minimo di democrazia reale. non si possono neanche regalare i miliardi a quello che è ormai, a tutti gli effetti, un regime, delegandolo a occuparsi dei profughi e a gestirne le sorti. È anche per queste ragioni che pensiamo che per l'Unione europea sia davvero un dovere politico e morale sospendere immediatamente l'accordo di cooperazione sull'immigrazione con la Turchia.

cordoglio per le vittime innocenti dei fatti che accadono in questo mondo sempre più drammatico, ma anche per ricordare ancora una volta che noi abbiamo il dovere, come Parlamento nazionale, di fare politica.

evidentemente hanno bisogno di un impegno straordinario e, ovviamente, di una quanto più larga possibile unità delle forze democratiche e progressiste di questo Paese e dell'intero Continente. Noi vogliamo fare fino in fondo la nostra parte e per questo crediamo

Signor Presidente, non sarò diplomatico. Questo tipo di commemorazione serve solo agli atti parlamentari. Il cordoglio ai caduti, ai feriti e al grande popolo francese, già provato da altri lutti, si è già espresso attraverso le parole del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio, alle quali il Gruppo di Area Popolare si associa convintamente. La veloce passerella di oggi pomeriggio sta riproponendo le posizioni di sempre delle forze politiche. Io spero che ci possa essere un passo avanti, un sussulto, cosa che dovrebbe avvenire in una Nazione civile e democratica, e la difesa del politicamente corretto e l'intensificazione dell'azione di vigilanza richiamate da chi sostiene invece il Governo. Lo sdegno per il massacro di Nizza spero non duri quanto quello di Dacca. E allora bisogna trovare le parole giuste, per capire ciò che sta accadendo dall'11 settembre 2001 ad oggi e che ha una più lontana origine nelle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 5 settembre 1972. Quarantaquattro anni in cui la risposta dei popoli arabi e islamici a presunti torti non è passata attraverso il confronto, il dialogo e la diplomazia, ma spesso attraverso le armi, le stragi, il terrore e comunque la morte straziante di innocenti. Bisogna trovare le parole e quelle giuste credo che coincidano con la definizione del fenomeno che ha dato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi: nazismo islamico. anni durante i quali si sono affermati etnie e popoli che, in virtù del loro islamismo o dell'interpretazione dell'islamismo, hanno commesso crimini nefandezze indicibili, dalla Nigeria alla Somalia, dall'Indonesia alle Filippine. Quarantaquattro anni nel corso dei quali molti hanno pensato che questo tipo di terrore fosse un fenomeno passeggero, che i principi della rivoluzione francese, dell'illuminismo, dell'emancipazione, della lotta al nazismo e al fascismo prendessero il sopravvento sulla barbarie terrorista ed estremista. L'Occidente e l'Europa in particolare hanno sperato che passasse la notte. E invece si è andata rafforzando la cultura dell'odio generata dal pensiero jihadista, cioè da un'interpretazione radicale dei versetti del Corano, non affatto contrastata dalle scuole coraniche. Le madrase in Italia sono circa un centinaio e questa interpretazione non la do io ma il vice presidente delle comunità musulmane francesi. Così la notte non passa e sangue innocente si aggiunge a sangue innocente. Dire che l'Islam non c'entra nulla è un gravissimo errore di sottovalutazione politica. Dire che non bisogna demonizzare l'Islam è solo una preposizione dialettica perché nessuno, in Occidente, in Europa e in Italia, ha posto problemi a questa pratica religiosa. Sperare che prendano il sopravvento le cosiddette aree moderate del mondo musulmano è parte di una politica suicida. Abbiamo sconfitto il terrorismo delle Brigate Rosse e dei NAR perché la nostra società ha isolato non le idee, che sono sempre rispettabili, ma l'uso della violenza per imporle. In questo caso non è così. Una parte consistente del mondo islamico potrà forse non condividere i metodi terroristici, ma non l'obiettivo di combattere gli infedeli che sono tali non solo perché sono crociati ma perché sono portatori di valori di democrazia, di laicità, di uguaglianza, di libertà e di parità tra i generi. Non si può chiedere solo alle Forze dell'ordine e ai servizi segreti di affrontare il terrorismo. Servono scelte unitarie, coraggiose, severe e ha fatto bene il Presidente del Consiglio a riunire ieri i Capigruppo di Camera e Senato. partire dall'isolamento e dal contrasto di quei Paesi islamici che foraggiano il terrorismo, altro che coprire le statue del Campidoglio per non turbare la sensibilità di un politico musulmano che non si turba, invece, quando nel suo Paese lapidano le presunte adultere, tagliano la testa con la scimitarra agli omosessuali e incarcerano e frustano a sangue chi difende i diritti civili. Il tutto perché in quel Paese, in quei Paesi, si rispettano alla lettera i precetti del Corano. Il realismo, direi il cinismo degli affari finanziari ed economici e la vendita di armamenti non può più essere accettabile per i Paesi democratici e quindi tra l'Europa e i sultanati, tra l'Occidente e i regimi totalitari, spietati e sanguinari. Presidente, mi avvio a concludere. nostro compito è difendere la sicurezza degli italiani, il futuro dei nostri figli ma anche le nostre conquiste di civiltà. Tra queste ritengo che la più importante sia quella dell'emancipazione femminile, spezzato le catene della tradizione, dell'ignoranza e della sottomissione maschile. In quest'Aula abbiamo parlato di tutto: dalla difesa degli animali agli OGM, abbiamo promosso commissioni d'inchiesta sugli argomenti e sui problemi più vari ma abbiamo ignorato che in Italia vivono decine, centinaia di migliaia di donne segregate, mantenute nell'ignoranza, sottomesse. Questo è il problema. Non è un problema secondario, è il problema perché l'Islam diventi una religione di pace.

le vittime in vittime sacrificali, state usando le persone come fossero cadute per la patria, cioè le state usando per i vostri scopi elettorali, per le vostre campagne elettorali. E ciò dal mio punto di vista è inaccettabile. Dico questo perché non dovremmo essere noi del Movimento 5 Stelle, che siamo gli ultimi arrivati, a dovervi ricordare come si fa e che cosa è una commemorazione. A me dispiace dover leggere i nomi dei sei italiani che nessuno di voi colleghi ha pronunciato. Voi avete parlato di Islam, di attacchi alla nostra civiltà. Ma quale civiltà? La nostra civiltà intesa come quella che professate voi? Perché nessuno di voi ha fatto i nomi dei nostri italiani? Non avete parlato assolutamente delle famiglie e del dolore che adesso sta accompagnando queste persone: le famiglie di Carla Gaveglio, Maria Grazia Ascoli, Gianna Muset, Angelo D'Agostino, Mario Casati, Nicolas Leslie. I nostri sei connazionali sono caduti a Nizza perché vittime di un terrorismo liquido,

sono caduti per un motivo fondamentale: non per i vostri rigurgiti tendenti al razzismo; sono state vittime e sono caduti perché hanno affidato le loro vite a noi a noi politici, e questo è un segno comune che hanno quei caduti con tanti altri caduti negli eventi che quotidianamente accadono non soltanto in in quei luoghi, ma in Italia e in tutto il mondo. Credo che la giusta commemorazione oggi andrebbe fatta non per un mero sperpero di campagna elettorale, come state facendo vergognosamente oggi pomeriggio voi; per

considerando il fatto che quelle persone vanno onorate, considerando questo momento come un punto di non ritorno. Dobbiamo dimostrare di aver compreso che d'ora innanzi il Governo e il Parlamento italiani, proprio per onorare loro e le loro famiglie, agiranno in un modo completamente diverso, ad esempio nella nostra politica estera, quindi non in maniera ipocrita, vendendo le armi con una mano e poi tendendo aiuti a quelle popolazioni con l'altra. Nessuno di voi si è chiesto: ma le armi utilizzate nelle stragi che avete menzionato, da quali Paesi arrivano? Arrivano per caso da Paesi con i quali noi facciamo affari? Nessuno di voi se lo chiede. allora con questa campagna elettorale. Dovremmo chiederci quanto quelle vittime e noi abbiamo in comune e condividiamo una politica estera fallimentare. Dobbiamo chiederci quanto di quello che è successo è imputabile anche alle nostre azioni. Questo significa essere un Governo e un Parlamento serio, maturo e responsabile. Ed è per questo che noi abbiamo chiesto che il Presidente del Senato e la Presidente della Camera convochino subito o siano di stimolo per una comunicazione del Governo in Assemblea, per riaprire il dibattito parlamentare su questi temi, perché lo riteniamo un passaggio fondamentale. Per questi motivi noi non accendiamo assolutamente la polemica sterile sulla visione politica di questi fatti, ma rimaniamo sul tema della giornata. Quindi il Movimento 5 Stelle esprime una vicinanza alle famiglie delle vittime. Con grande cordoglio e con grande 5 Stelle all'interno del Parlamento è pronto ad avviare una fase nuova di dibattito e di discussione proprio per onorare le vittime e le famiglie di Nizza.

alle famiglie colpite da questo ennesimo episodio di terrorismo. Mi riferisco alle famiglie dei francesi ma anche degli italiani presenti a Nizza, che dopo vari giorni faticosamente sono stati identificati, nell'angoscia ulteriore delle loro famiglie che per giorni hanno atteso, alimentando la labile speranza che i loro cari non fossero sulla Promenade des La tragedia quindi colpisce il popolo francese, ma anche la nostra Nazione, non solo per le nostre vittime, ma anche perché Nizza, la città dove nacque Garibaldi, è un incrocio di storie, di passioni, di civiltà e di culture che legano intimamente l'Italia e la Francia.

E la sera dopo accade una vicenda diversa, lontana, ma poi non troppo, da questa che stiamo oggi commemorando. La vicenda della Turchia, che ci ha lasciato ancora di più disorientati e ci ha fatto capire, colleghi, che noi stiamo vivendo un momento drammatico. È stato il Santo Padre, e non un'autorità politica di parte, a dire qualche mese fa che noi stiamo vivendo una terza guerra mondiale che viene combattuta a pezzi. Purtroppo, l'affermazione del Santo Padre, uomo di pace e di solidarietà forse ancor più dei suoi predecessori, ha richiamato al realismo tutti noi. È una guerra che si combatte con l'instabilità della Turchia,

scossi da eventi che non possiamo che definire di natura bellica. Noi siamo quindi di fronte a una tragedia che si può rinnovare in qualsiasi momento, viste anche le circostanze della vicenda di Nizza, con il camion che trasportava i gelati (ovviamente inesistenti) da consegnare e, forse, anche sicurezza della Francia, appena uscita dagli Europei di calcio, un appuntamento cui si guardava non solo per lo sport ma anche per la preoccupazione che il terrorismo potesse cogliere quella occasione anche di festa popolare e di gente radunata, non solo nelle città della Francia ma in tutta Europa davanti a uno schermo. Ebbene, forse questo intervenire quella sera ha voluto richiamarci, con un realismo che, purtroppo, dobbiamo ormai consapevolmente nutrire tutti noi, al fatto che il terrorismo può colpire ovunque e comunque.

Ieri sera in Germania un altro lupo solitario, un diciassettenne afgano, ha colpito in un treno. La persona che ha colpito a Nizza era forse un altro lupo solitario, ma entrambi non sono estranei alla radicalizzazione del fondamentalismo islamico. L'ISIS li proclama propri soldati, ed è quindi inutile andare a fare l'analisi della connessione maggiore o minore. Perché una connessione c'è: quella di un fanatismo ideologico, di un grande califfato che si vuole espandere. Allora il Governo italiano non deve solo incrementare le misure di sicurezza.

Noi non siamo immuni da tutto quello che sta accadendo. Servono leggi di natura eccezionale da concordare a livello globale. Servono misure adeguate di controllo. Forse dobbiamo anche cambiare le nostre abitudini abitudini di vita, come le cambiammo nelle stagioni drammatiche del terrorismo interno in Italia, assumendo cautele e controlli che un tempo non esistevano. Ma sottovalutare la portata ideologica,

l'arma del dialogo? Ma l'attacco alla nostra civiltà, alla nostra cultura e alla nostra convivenza c'è. E anche il fatto di avere integrato persone che hanno trovato lavoro e accoglienza nei nostri Stati, come accade in Italia ed è accaduto anche in Francia, ebbene, a volte non ha scaturissero dalle menti perverse di alcune di loro questo fanatismo e questa predicazione. Non temiamo accuse di razzismo e riteniamo che i valori costituzionali dell'Italia e della Francia vadano salvaguardati, ma abbassare la guardia e non rendersi conto che siamo dentro una guerra - come, lo ripeto, ha detto persino l'uomo più di pace del

Signor Presidente, colleghe e colleghi, abbiamo avuto in quest'Aula, negli ultimi tempi, tante occasioni di manifestare cordoglio e solidarietà. Questa volta sentiamo che il colpo è stato più forte, più profondo. Per l'efferata dinamica dell'attacco o perché tra le vittime innocenti si annoverano molti bambini. Le immagini spezzano davvero il cuore, A nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico ripetiamo allora con più forza, con la determinazione che viene da un dolore più profondo e lancinante di sempre, la nostra condanna e la nostra vicinanza ai familiari delle vittime, alla città di Nizza, al popolo francese. La strage è di tale barbarie che porta, almeno me, a collocare in secondo piano il tempo delle analisi e delle valutazioni politiche e strategiche. Sarà sicuramente necessario farle, e bene, in sedi e momenti appropriati. Spero che tutti vi partecipino attivamente, anche chi finora si è sottratto all'impegno comune. Ma intanto bisogna porci pienamente dalla parte delle vittime. Le parole che più frequentemente definiscono la strage di Nizza sono orrore, crudeltà e assurdità. Le ritroviamo nella lettera inviata da tutti i Capigruppo del Senato all'ambasciatrice di Francia a Roma, che saluto con grande rispetto: iniziativa giusta e lodevole. Queste terribili parole non possono risuonare solo per pochi giorni ed essere poi sostituite dai contrasti sul come fronteggiare il terrorismo. Esse debbono scuotere la nostra coscienza morale e ispirare le nostre azioni. Non indugerò dunque sui commenti o sulle dispute già in corso. Mi limito a qualche breve annotazione, preliminare alla discussione che faremo. La prima è che l'abisso culturale ed esistenziale in cui il terrorismo vuole condurci è l'esatto opposto dell'immagine di vita e di socialità che esprimevano i tanti presenti a Nizza il 14 luglio. Ad un umanesimo di valori, di partecipazione e di convivenza (pur con tutte le sue contraddizioni) si è contrapposta la barbarie dell'odio e dell'annientamento di chi ha idee e credo diversi. È giusto gettare l'allarme per questa sconvolgente deriva. Violenza e terrore si possono vincere, e io penso che li vinceremo, con la fermezza e con l'intelligenza. Ma il prezzo sociale e culturale sarà pesante e duraturo, in termini di arretramento delle possibilità e della qualità del dialogo, dello scambio culturale, della cooperazione umana. La trappola dell'imbarbarimento è davanti a noi, spalancata e tentatrice. Credo che in nome di chi è morto a Nizza dobbiamo evitare di caderci. un pensiero speciale va al popolo francese, alle sue istituzioni, alla sua cultura e storia. Il terrorismo jihadista ha colpito più volte quel Paese, cercando di sfregiare il messaggio universale che tutti riconosciamo nel motto *egalité, liberté, fraternité*. Sentirsi vicini alla Francia vuol dire, però, capire il suo dramma terribile: il rischio, cioè, di una guerra civile vera, che incendi città e periferie. Se dovesse essere così - sappiamolo - la cosa non si fermerà alla Francia. Potremmo essere coinvolti tutti. Per questo dobbiamo aiutare i francesi a vincere il mostro dell'intolleranza e della violenza. da Nizza arriva la chiamata ad una visione alta, matura e consapevole della politica. Rispetto alla gravità del momento colpisce la modestia e l'inadeguatezza di molte delle battaglie o delle scaramucce di casa nostra. Nell'attacco all'Europa c'è anche una sfida alla sua indebolita cultura politica, alle crescenti difficoltà di misurarsi con fenomeni nuovi e dirompenti. Occorre seriamente lavorare, da tutte le sponde politiche, senza eccezione alcuna, per un salto vero della nostra cultura politica. La stessa ripetitiva discussione sulle colpe del buonismo o del muscolarismo

quello di non farci trascinare nel gorgo dell'impotenza e dell'irrilevanza, per omissione o per incapacità di capire, di pensare e agire in modo nuovo. Questo per me vuol dire mettersi dalla parte delle vittime. Da lì si parte per vincere la sfida.

ci associamo alle sue parole, che condividiamo con spirito sincero, e siamo naturalmente vicini alle famiglie delle vittime italiane. però, non distinguiamo tra morti italiani, morti francesi, morti americani, morti armeni, morti russi, morti ucraini.

le rinnovo i sentimenti di profonda vicinanza e amicizia già trasmessi al popolo francese dal Presidente della Repubblica. È stata colpita la Francia, ma ad essere colpiti siamo stati tutti noi. Non è, signora ambasciatrice, un *tweet*, ma la consapevolezza che ad essere sfregiato è chiunque si richiami ai valori civili e inclusivi della Rivoluzione francese. Non a caso, proprio nel suo Paese si colpisce di più; si colpisce di più laddove i valori più profondi hanno plasmato il mondo moderno, e l'integrazione non è un disvalore, è davvero un prodotto di quei valori. La paura che rischia di entrare in noi, che è già in noi, ha l'obiettivo, appunto, di colpire quei valori ed è l'obiettivo vero dei terroristi, per scatenare lo scontro tra civiltà; ma il tema non è lo scontro tra civiltà, con un uso, da parte del terrorismo, fanatico, strumentale delle religioni. A questo noi non possiamo acconciarci. La nostra libertà non può essere contenuta nel filo spinato. Pertanto, integrazione e legalità devono camminare insieme senza schizofrenie: lo chiediamo al Governo turco e lo dobbiamo praticare noi. La solidarietà e la costruzione europea devono essere le prime risposte; non lo scontro tra

dal Santo Padre. Non i muri infrastatali, ma la frontiera europea è la strada da perseguire per combattere il terrorismo. Più Europa dunque e non meno Europa: l'Europa dei valori e l'Europa dell'*intelligence*, l'Europa degli scambi e l'Europa dei controlli. A questo siamo saldamente ancorati oltre ogni strumentalità e io penso che le polemiche strumentali debbano lasciare il campo alla consapevolezza del momento in cui siamo e delle risposte che insieme siamo chiamati a dare. A questo fine immagino la seduta delle Commissioni esteri di Camera e Senato, già programmata per la prossima settimana nella giornata di martedì, e spero che in quella occasione Parlamento e Governo insieme sapranno offrire il meglio delle culture democratiche.

Proprio perché queste parole sono importanti, il dibattito si è svolto secondo le varie sfumature di ogni Gruppo parlamentare, secondo quello che ognuno di noi rappresenta, dando conto dell'idea che ogni cittadino italiano ha di quello che è successo e di quello che sta succedendo. Proprio per questo motivo vorrei

Gruppo LN-Aut)*. Signor Presidente, siamo in un momento storico importante, drammatico, in cui sono stati uccisi cittadini francesi e italiani, in cui

quello che sta succedendo e che è successo poche ore fa in Francia, dove un marocchino ha aggredito una mamma con tre bambine, ferendo gravemente una di queste. Potrei andare avanti: a Trento le Forze dell'ordine sono state la denuncia - arrivata in questi giorni - secondo cui nel 2015 più di 1.000 poliziotti sono stati aggrediti nell'esercizio delle loro funzioni e proprio oggi i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei militari e dei carabinieri ci dicono di non avere i mezzi per difendersi e per poter tutelare la sicurezza dei cittadini.

non punisce il reato di tortura, ma limita l'operato delle Forze dell'ordine. Lo abbiamo sentito anche in quest'Aula: finalmente la polizia non potrà più fare quello che vuole.

I sindacati di polizia chiedono il ritiro di questo provvedimento; il capo della polizia l'ha criticato; il ministro Alfano, una volta tanto, con un atto di dignità uno, finalmente: un atto di dignità nel suo periodo da Ministro dell'interno - ha detto che forse questo provvedimento non va bene così com'è. Ma tanto si andrà alla Camera a modificarlo, signor Presidente. se c'è il bicameralismo prefetto - chiedo a voi sapientoni della Costituzione - perché non lo modifichiamo già in questa sede, facendo vedere che il Senato è in grado di lavorare?

quanto sia stato tormentato il percorso di questo provvedimento, quante criticità abbia evidenziato anche all'interno dei Gruppi che hanno discusso di questo tema. Il fatto nuovo rispetto alla discussione che è avvenuta questa settimana è rappresentato innanzitutto dalla presa d'atto di un problema da parte del Ministro dell'interno in una sede istituzionale: eravamo a Palazzo Chigi, Grazie la rappresentazione simbolica dell'unità del Paese rispetto a un'emergenza, in questo caso, di terrorismo e di sicurezza per il Paese stesso. A fronte di quanto noi di Forza Italia abbiamo detto rispetto a questo provvedimento, il Ministro dell'interno ha preso atto della problematicità

penso che la richiesta del collega Centinaio sia quanto mai opportuna. Infatti, al di là del merito del disegno di legge, che che offre riflessioni importanti, tanto quanto quelle sulla tutela delle nostre forze di polizia, è chiaro a tutti che è intervenuto un evento che, ancora di più, pone all'attenzione di tutti noi il problema di capire se, all'interno di quel disegno di legge,

intervenuto poi in Assemblea a modificare quel testo? È intervenuto un fatto che tutti abbiamo considerato sbagliato. Come ci dimostrano le proteste serie e vibranti delle forze di polizia e sicurezza, quel testo ha tradito

quindi ben volentieri alla proposta del collega Centinaio ma chiedo di fare di più. Non ci si nasconda dietro al fatto che oggi la Conferenza dei Capigruppo - che sono certa lei convocherà seduta stante - rinvierà a chissà quando e dove l'esame del provvedimento, perché questo è un alibi comodo che serve a chi

ma rimediarvi attraverso il ruolo di legislatori responsabili. In un frangente come questo ci è richiesto di essere innanzitutto protagonisti della nostra missione, cioè quella di rappresentare i cittadini e di legiferare interesse, e nell'interesse dei cittadini italiani il rispetto delle forze di polizia e di sicurezza non può mai essere messo Quando accadono fatti per i quali le responsabilità personali di ciascuno sono chiamate in causa, la risposta della legge e di tutti noi deve essere chiara e ferma, contro Questo non vuol dire, con la scorciatoia adoperata dal Partito Democratico e da chi ha proposto quell'emendamento,

anche nei confronti dell'ordinamento giudiziario, che dovrebbe confermare e sostenere lo sforzo che le forze di polizia compiono ogni giorno; accade invece che talvolta talvolta quelle stesse forze abbiano l'impressione di lavorare su una tela di Penelope: loro la fanno e qualcun altro la disfa.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di posporre l'esame del disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura al fine di un ulteriore approfondimento del testo. Questa sera, dopo le decisioni sul calendario dei lavori, l'Assemblea passerà alla deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione. Nella seduta antimeridiana di domani saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e inizierà l'esame del disegno di legge di delegazione europea. Nella seduta pomeridiana, con inizio alle ore 16, saranno esaminati il rendiconto e il bilancio interno del Senato. La discussione si concluderà entro domani sera. Gli ordini del giorno dovranno essere presentati entro le ore 11 di domani. Nella seduta antimeridiana di giovedì 21 luglio, proseguirà la discussione sulla legge di delegazione europea, auspicabilmente fino alla sua conclusione. Nella seduta pomeridiana di martedì 26 luglio sarà posto all'ordine del giorno il decreto-legge sulla cessione dell'ILVA di Taranto. Nel corso della prossima settimana sarà nuovamente convocata la Conferenza dei Capigruppo, per definire l'ordine, ferma restando la priorità dei decreti-legge in arrivo dalla Camera,

Presidente, noi riteniamo assolutamente grave la decisione presa e la proposta

Io trovo incredibilmente vergognoso il fatto che, dopo la commemorazione delle vittime di Nizza, si siano utilizzati strumentalmente quei morti per compiere l'operazione, cui si ambisce ormai da molto tempo, di bloccare il disegno di legge sulla tortura. con motivazioni che già nel merito, la scorsa settimana, avevamo - a mio avviso - puntualmente e in modo inoppugnabile contestato. Si fa una rappresentazione di quel disegno di legge, e anche della decisione assunta da quest'Aula

ha detto assolutamente nulla e ha lasciato tutto ai commenti e alle indicazioni del Ministro dell'interno, che ieri si è permesso

perché si sta interferendo con l'attività parlamentare e questo - torno a ripetere - è un cedimento a una strumentalità vergognosa, tanto più che ciò è avvenuto dopo gli interventi di commemorazione dei morti e delle vittime di Nizza. Lo trovo veramente incredibile.

essere più forti nel combattere il terrorismo e non strumentalizzarlo per abdicare al nostro dovere. Cosa dobbiamo dire? Che hanno vinto loro? Perché questo significa fare in modo che possano vincere loro e questo noi non lo permetteremo.

Mi soffermo però sul provvedimento sulla tortura e vorrei brevemente rimanere nel merito di quel provvedimento chiarire che nelle intenzioni del nostro Gruppo non c'è assolutamente collegamento tra questa preannunciata sospensione di Nizza che abbiamo discusso e affrontato all'inizio di questa seduta pomeridiana. Su questo provvedimento sono state sollevate diverse, interessanti e importanti questioni. Questo provvedimento - com'è stato già detto - si trascina da oltre una ventina di anni. Le questioni sollevate erano tutte protese a distinguere la tortura da altre tipologie di reati che risultano già contestati,

più violenze, più minacce e per noi quindi incorpora il «reiterato». A tal riguardo è stata fatta un'obiezione e cioè che l'eliminazione del «reiterato» possa ingenerare la confusione che si voleva, appunto, eliminare. Noi pensiamo che l'uso del plurale sia in sé sufficiente, ma proprio questa convinzione ci ha portati a richiedere nella sede dei Capigruppo un'ulteriore riflessione su un provvedimento che è da tanto tempo in discussione. Una sospensione, non un binario morto; una sospensione che sia dinamica, che possa produrre frutti e si ponga l'obiettivo di raggiungere in quest'Assemblea un'ampia convergenza delle forze parlamentari.

sul fatto che debbano essere tutelate e difese le Forze dell'ordine nel momento in cui difendono il nostro stato di diritto, nel momento in cui si sacrificano per far rispettare le leggi. Come ho detto, siamo stati noi a sostenere che fosse data la possibilità di un'ulteriore riflessione, quindi una sospensione breve - ma non definitiva - del disegno di legge. Con questo vorremmo eliminare ogni strumentalizzazione, ogni ombra, ogni sospetto, perché riteniamo che questo provvedimento meriti il consenso di tutta l'Assemblea.

veramente tutto il possibile perché il provvedimento sulla tortura torni nell'Assemblea del Senato per essere approvato prima dell'inizio delle ferie estive. Ripeto quanto detto. L'Italia ha un debito molto alto con i suoi cittadini, con le Forze dell'ordine e con la comunità internazionale per un ritardo che ormai supera le tre legislature. È un provvedimento che non intendiamo abbandonare. Abbiamo accettato - debbo dire non volentieri - la sospensione, perché riteniamo riteniamo essenziali due elementi che vanno in ogni modo salvaguardati: anzitutto, dobbiamo avere la certezza di una maggioranza che approvi il provvedimento; dopodiché, vogliamo che questa maggioranza sia molto ampia. Poco fa in Conferenza dei Capigruppo ho fatto un appello a tutti i Capigruppo

Non è così, come sapete. È un provvedimento che riguarda chiunque; è una norma applicata a qualunque cittadino dovesse commettere il reato che è stato ipotizzato e definito

Presidente, la legge sull'introduzione del reato di tortura nel nostro Paese è un atto dovuto ed è di una gravità inaudita che questo Parlamento nazionale per tanti anni non abbia ottemperato a quello che era un obbligo internazionale,

una cosa che invece avrebbe dovuto vedere unito questo Parlamento e questo Paese, le sue forze democratiche e progressiste. Noi consideriamo del tutto inaccettabile che venga utilizzata la drammatica situazione internazionale per mettere in secondo piano questo provvedimento e lo riteniamo ancora più inaccettabile oggi. Presidente Zanda, glielo voglio dire con grande nettezza: oggi è il 19 luglio 2016

Per me che a Genova 2001 c'ero e che ho ancora addosso quella ferita indelebile, la vicenda di oggi e questo rinvio *sine die* dell'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano è veramente qualcosa senza precedenti, molto più grave di tanti altri provvedimenti, pure sbagliati,

non avevamo bisogno dei fatti di Nizza per appoggiare una proposta di buon senso, quella cioè di prendere una pausa di riflessione e di approfondimento su questo provvedimento. Signor Presidente, il Parlamento non si deve far condizionare da fatti esterni, ma non può essere nemmeno in una torre eburnea nella quale non arrivano gli echi di quanto accade fuori e in questi giorni ho l'impressione che siano accadute due cose

che i sindacati di polizia, dei quali si era dubitato avessero una posizione uniforme, l'hanno invece confermata e lo hanno fatto manifestando in maniera pubblica

deve essere registrato e diventa un fatto politico che merita una risposta. In secondo luogo, ho letto un'intervista del Ministro dell'interno nella quale si ipotizza la possibilità che le Forze dell'ordine rimangano armate anche fuori dal loro orario di lavoro. È evidente che una misura del genere, qualora dovesse essere soltanto ipotizzata,

la nostra perplessità è forte e in qualche modo è questo il punto che chiede di essere approfondito.

che, invece, deve essere tenuta in conto. Questo provvedimento non riesce a fissare il limite tra l'abuso dell'uso legittimo della forza e la tortura. Per questo, senatore Zanda, i nostri dubbi fanno riferimento soprattutto alla relazione che le Forze dell'ordine hanno con questo provvedimento. È evidente che il reato parla a tutti e non solo alle Forze dell'ordine, ma solo per le Forze dell'ordine c'è questo problema specifico: dove passa il confine tra l'abuso di un uso legittimo della forza - che non è tortura e il reato di tortura? Nessuno di noi dubita che il reato di tortura abbia la possibilità di essere preso in considerazione e di essere introdotto. Da questo punto di vista, vale la proposta fatta dal senatore Giovanardi, se volete, in modo in modo esemplare: prendiamo il testo della Convenzione di New York e facciamolo diventare legge. Questo per dire che nessuno ha un'opposizione all'introduzione di questo reato in generale; ma il testo che ci è stato consegnato non riesce a dare garanzie alle Forze dell'ordine.

potrebbe presentarsi troppo tardi rispetto allo sconvolgimento che un'accusa specifica può portare nella vita di un servitore dello Stato onesto, che non sa e non riesce a cogliere qual è il punto di discrimine. Noi, quindi, accogliamo positivamente la decisione della Conferenza dei Capigruppo, ma vorremmo che non si trattasse di un'ipocrisia. Vorremmo che questa sospensione fosse legata alla volontà politica di un approfondimento serio e di un provvedimento garantista nei confronti dei servitori dello Stato, che riesca a chiarire loro - e quindi anche a noi dove passa il confine tra quanto è lecito e quanto non è lecito e tra quanto non è lecito e quanto è tortura; perché non tutto ciò che non è lecito può essere definito tortura. Questi sono i quesiti seri e strutturali che rimangono in capo a questo provvedimento e ai quali chiediamo risposta. Pertanto, o la sospensione serve a questo o serve a passare la nottata e a collocare il provvedimento in esame in un contesto mediatico migliore, ma

quindi al mittente certe affermazioni offensive. Faremo di tutto, cari colleghi, affinché questo provvedimento rimanga in coda all'ordine del giorno. Abbiamo fatto di tutto oggi, abbiamo fatto di tutto durante la Conferenza dei Capigruppo e faremo di tutto affinché questo provvedimento non venga trattato o venga trattato il più tardi possibile.

Non è colpa mia se qualche giorno fa a Nizza è successo quello che tutti sappiamo; non è colpa mia se quotidianamente in Italia succedono atti di violenza. Di conseguenza, non è colpa mia se oggi, dopo la trattazione

Dobbiamo approvare modifiche al calendario dei lavori. Ringrazio per gli interventi *ad adiuvandum*. Se così sono, che siano brevi. Ne

atteso da oltre ventiquattro anni, in questo clima di contrasto sicuramente non fa onore a questo Parlamento. Il provvedimento dovrà essere calibrato in modo da assicurare la doverosa tutela dei cittadini con la copertura normativa delle necessarie operatività dei tutori dell'ordine. L'intervento di mediazione

che vadano a mettere delle toppe dove noi abbiamo lasciato dei vuoti. Questo è il nostro dovere di legislatori: fare in modo che il provvedimento venga licenziato in maniera chiara. Senatore Zanda, non insista con quel plurale comparabile all'eliminazione del termine «reiterate». Andiamo avanti, superiamo l'ostacolo e cerchiamo di trovare una formula

sottoposto alla custodia delle Forze dell'ordine dovrebbe essere più sicuro che a casa propria. Francamente, mi sento di difendere le Forze dell'ordine

La mia proposta, Presidente, visto che i tre obiettivi sono condivisi da tutti, è di tornare in Commissione e di sistemare questa norma esattamente come la Convenzione di New York ci chiede di fare. Leggete la Convenzione di New York e vedete cosa si intende lì per tortura. Io sono perfettamente d'accordo con la Convenzione di New York,

a me pare la più rispettosa del ruolo di questo Parlamento e della Commissione, la quale - giusto per ricordare come sono andate le cose - aveva esitato un testo che raccoglieva il massimo consenso della rappresentanza di questo Parlamento.

Grazie

che penso non interpreti la stragrande maggioranza di quest'Assemblea, divisa in una tifoseria che non c'è.

il nostro Paese è in grande ritardo (quindi deve poterlo fare). E si deve ricordare che quel reato non è riconducibile in prima istanza alle nostre forze di polizia e sicurezza; lo ha già detto bene prima il collega Quagliariello e non mi ripeto.

rispondano del reato che commettono. Se su questo tema c'è l'esigenza, come mi pare, di una serena discussione, il testo deve tornare in Commissione, perché solo la Commissione ha la capacità, le competenze e lo lasci ricordare, signor Presidente - il ruolo per svolgere questo lavoro. Non ce l'hanno i Capigruppo, secondo me, signor Presidente; i Capigruppo svolgono un'altra funzione. In questo caso, la prego di non esautorare la Commissione dal suo ruolo, perché lei in questo modo

Le posso anche dimostrare il motivo per cui faccio questa affermazione; con grande convinzione e rammarico, certo, ma anche con la convinzione di chi lo può dimostrare. Moltissimi, quasi tutti gli interventi che si sono succeduti si sono soffermati sull'eliminazione del termine «reiterate». Nel merito, come può pretendersi

prima di me. Sarebbe giusto e corretto fare l'elenco di tutti i 231 nomi. Invito i rappresentanti delle Forze dell'ordine a farlo. Io l'ho fatto: è agli atti.

che mancano i protocolli operativi per le Forze dell'ordine, protocolli che siano rigorosi, dettagliati ed efficaci. Di questo c'è veramente bisogno per tutelare le Forze dell'ordine nel nostro Paese.

chiesto e auspicato nella seduta di oggi. Voglio ricordare, a chi parla di strumentalizzazioni, che noi avevamo già espresso giovedì i nostri dubbi su questa stesura del testo, quindi indipendentemente dagli eventi drammatici che hanno sconvolto l'Europa

non contenevano la parola «reiterate» ma limitavano la configurazione di questo ipotetico reato, evitando, ad esempio, che l'attività istituzionale che viene svolta (penso ad una manifestazione di piazza) potesse essere configurata come occasione di tortura. Noi rivendichiamo il merito di questa pausa di riflessione e verificheremo

Prego

Molti di noi sono sempre stati presenti in quel luogo; oggi siamo qui a lavorare e vogliamo ricordare anche da quest'Aula il 19 luglio di ventiquattro quando la storia del nostro Paese fu sconvolta dall'ennesima strage di mafia, la strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino

Il nostro Paese non si rassegna, non si deve rassegnare. È una storia che ancora oggi deve parlare alla coscienza di tutti. E così è in molte scuole, nelle nuove generazioni. Deve continuare a interrogare i rappresentanti delle istituzioni e fare in modo che si continui a ricercare la verità, tutta la verità. Molti ritengono che questa sia una *mission impossible*, perché intorno alle stragi il sistema delle collusioni spesso impedisce che si possa giungere alle più amare e terribili verità. Ma quelle amare e terribili verità sono in grado di spiegare perché nel nostro Paese,

della trattativa avviata con cosa nostra, con in testa Totò Riina. Era anche rammaricato di quel modo di presentare la sua candidatura alla procura nazionale antimafia. Rammaricato, arrabbiato e amareggiato, perché sentiva in quella candidatura il tratto dell'isolamento e non della responsabilità di guidare una importante istituzione, pensata e voluta da Giovanni Falcone. amareggiato della mancata protezione, come si ricava da una lettura attenta e onesta di quei giorni. Una mancata protezione che lo ha esposto anche quando si recava a casa della madre. E così anche dalla sottrazione dell'agenda rossa, quell'agenda in cui egli segnava i suoi pensieri, le responsabilità il sistema delle collusioni. Ecco perché, signor Presidente, non dobbiamo rinunciare alla ricerca della verità, naturalmente con diversi strumenti: quelli giudiziari, che spettano alla magistratura,

Spetta alla democrazia, nel nostro contesto parlamentare, visti i poteri della Commissione, andare sino in fondo e non sottrarsi alla ricerca Presidente, quelle stragi, come lei ha potuto vivere anche da protagonista, hanno segnato la storia del nostro Paese. Dobbiamo fare in modo che la storia che insieme dobbiamo costruire sappia fare memoria, raccontare i fatti come sono andati e fare in modo che nel nostro Paese le mafie siano battute e eliminate dal

Una persona che ha lottato per la legalità e contro la criminalità con il sentimento di servire lo Stato, con il sentimento di servire la gente attraverso un'azione un'azione di giustizia. Un uomo che ha messo se stesso molto dopo l'adempimento del proprio dovere, perché sapeva ogni giorno di rischiare la vita. ha perso. Direi che egli è stato un esempio sotto ogni punto di vista, non solo nell'ambito della lotta alla mafia, che va perseguita con determinazione, ma in generale per tutti coloro che servono lo Stato e per tutti i cittadini del nostro Paese.

fervido di quei due servitori dello Stato che sono stati Falcone e Borsellino. E lo ero quando Falcone e Borsellino erano duramente contestati dentro la magistratura (e non solo) ed erano stati fatti anche oggetto di campagne denigratorie e calunniose nei loro confronti. Hanno perso la vita perché combattevano la mafia. Chi ha letto il famoso libro di Giovanni Falcone o ha ascoltato ciò che diceva Borsellino, sa che essi teorizzavano che, come tutte le vicende umane, la mafia poteva avere un inizio, uno svolgimento e una fine. Quindi la mafia poteva essere piegata, ma la mafia ma la mafia approfittava delle collusioni che poteva trovare dappertutto per alimentare il suo potere. Falcone non correva dietro ai teoremi politici, Falcone combatteva i mafiosi duramente, sapendo anche distinguere la realtà dei pentiti veri da quelli che invece erano calunniatori e volevano depistare. Allora, collega Lumia, mi associo al primo passaggio del suo intervento e sono d'accordissimo

PD)*. Su questo non sono d'accordo perché credo che lo Stato ci sia, con i magistrati, con il Governo

Signor Presidente, ringrazio il collega Lumia per averci voluto ricordare in chiusura d'Aula una giornata così importante. E siamo ben poca cosa noi tutti, senatore Lumia, lei, io, forse persino il presidente Grasso che pure con quella stagione, con quegli uomini, ha lavorato e quella legge e quella patria ha servito. Siamo ben poca cosa anche rispetto a quella retorica dell'antimafia che ha finito per farci sembrare una giornata come questa una giornata come le altre, quando invece non è così. è così. Oggi, come ogni giorno, come domani, come dopodomani; e rivolgo questo accorato appello al presidente Grasso, che è al tempo stesso senatore tra i senatori, Presidente del Senato, e uomo di legge, affinché il ricordo non sia limitato a questo e sia invece l'occasione per riflettere, come sempre dovremmo fare e come sempre ci sforziamo di fare, in ogni provvedimento che votiamo, sul significato che ha avuto nella storia del nostro Paese il sacrificio di quei due uomini e prima di loro di molti altri: magistrati che hanno pagato con la vita servire lo Stato,

(da una parte chi difende una cosa e dall'altra chi ne difende un'altra), penso che questo ricordo - che auspico possa essere una celebrazione più importante di quella poca cosa che stiamo facendo qui oggi e in questo momento - ci aiuti a distinguere quel bene supremo al quale tutti tendiamo - ne sono certa pur rispondendo a visioni politiche della società diverse che possono farci sembrare divisi. Ma sono certa che nel ricordo di un uomo e dei tanti uomini come lui e delle molte donne che in quell'ambito e non solo sacrificano e dedicano la loro vita a servire questo Paese, in quel ricordo oggi dobbiamo trovare la forza per non smentire il ruolo di questo Parlamento. allora, un appello a lei, signor Presidente, perché sia il nostro garante, come lo è sempre, anche di una celebrazione che non è solo quella della memoria, ma è quella dell'impegno quotidiano. La ringrazio per quanto vorrà fare per fare sembrare meno piccolo di noi, di me o del senatore Lumia, il ricordo di questa giornata.

Paolo Borsellino lascia un'eredità di valori, un patrimonio morale che non si dovrà mai disperdere. Quest'Assemblea e ciascuno di noi dovrà contribuire a perpetuarne la memoria. Ringrazio comunque per questo momento, che mi fa sentire parte di un'Assemblea che sente ancora questi valori e li vuole perpetuare. *(Applausi)*.

con questo intervento di fine seduta prosegue, oggi, una staffetta con cui, assieme a tante altre senatrici e a tanti altri senatori, ricorderemo ogni donna che verrà uccisa per mano di un uomo, a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. Il marito l'ha ammazzata in casa, con almeno tre martellate alla testa; l'avrebbe poi strozzata e si è subito costituito, ha confessato. Era l'alba di sabato, l'abitazione, una villetta in provincia di Varese, a Laveno Mombello, è stata subito raggiunta dal 118, ma non c'era più nulla da fare: Loretta Gisotti - questo il nome della donna - cinquantaquattro anni, una *make-up artist* diplomata, era già deceduta per le gravissime ferite inferte. Tensione tra i due coniugi in partenza per le vacanze: motivi banali, pare. Ma un femminicidio al giorno sembra non bastare. A Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, i carabinieri hanno fermato, sempre nella notte tra venerdì e sabato, Giovanni Baiada, ottant'anni, pensionato, con l'accusa di avere ucciso la moglie, Maria Licari, settant'anni, con un colpo alla testa. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Palermo. Secondo quanto ricostruito dai militari, il fatto sarebbe accaduto nel corso dell'ennesima lite. L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni una donna viene uccisa. Il 46,3 per cento di queste donne muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita. La violenza sulle donne è quasi sempre descritta come frutto di motivi passionali. Lo stereotipo dell'onore tradito, che giustificava il delitto d'onore, si trasforma in quello della gelosia, del tradimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. Il *partner* sarebbe, quindi, un soggetto da compassionare per essersi lasciato trascinare ad un gesto estremo (un *raptus*, magari). Una spiegazione, insomma, che, dando una attenuante al colpevole, addosserebbe alla donna una parte di responsabilità, perché in qualche modo responsabile di avere suscitato la gelosia. Si tratta di una falsa rappresentazione della realtà. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data, spesso non denunciati. Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che affonda le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomini e donne. Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne e nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna, però, monitorare che queste misure

e soprattutto si dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Un appello al Paese: sono 160 le donne uccise ogni anno, non possiamo più accettare questa mattanza. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, ha designato il 25 novembre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Noi vogliamo celebrare questa giornata ad ogni femminicidio.

La seduta è tolta